La Conferenza dei Capigruppo ha definito il nuovo calendario dei lavori. Nella seduta di oggi il Presidente renderà le comunicazioni, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, sul disegno di legge di bilancio, propedeutiche all'assegnazione del provvedimento che darà inizio alla sessione di bilancio. La 5a Commissione permanente dovrà concludere i propri lavori entro le ore 13,30 di domani. Conseguentemente, i rapporti delle Commissioni permanenti dovranno essere trasmessi in tempo utile. Gli emendamenti per l'Assemblea dovranno essere presentati entro il termine di un'ora rispetto a quello fissato in Commissione. quindi alla discussione del decreto-legge sul rilancio del servizio sanitario della Regione Calabria. Poiché il Governo ha preannunciato l'intenzione di porre la questione di fiducia, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che la discussione sulla fiducia sia ricompresa nella discussione generale del provvedimento. Quest'ultima si svolgerà, fino alla sua conclusione, nella seduta di oggi, che non prevede orario di chiusura. Domani, alle ore 9,30, avranno luogo le repliche del relatore e del Governo, la votazione del non passaggio agli articoli preannunciata dal Gruppo Forza Italia, le dichiarazioni di voto e la chiama. Dopo il voto di fiducia sul decreto-legge, intorno alle ore 13,30 avrà inizio la discussione del disegno di legge di bilancio, secondo le seguenti scansioni temporali. Per la discussione generale sono state ripartite sei ore e trentacinque minuti in base alle richieste dei Gruppi. Seguirà la replica del Governo. Conclusa tale fase procedurale, si passerà al voto degli articoli della seconda sezione del disegno di legge di bilancio (e di eventuali emendamenti). Tali votazioni hanno la precedenza sull'esame della prima sezione (articolo 1), ai sensi dell'articolo 129 del Regolamento. Poiché il Governo ha preannunciato l'intenzione di porre la questione di fiducia sull'articolo 1, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, la Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione della relativa discussione. Per la discussione sulla fiducia, che avrà inizio mercoledì 30 dicembre, alle ore 9, sono stati ripartiti un'ora e trenta minuti in base a specifiche richieste dei Gruppi. Seguiranno le dichiarazioni di voto e la chiama. A conclusione della chiama si passerà al voto finale elettronico del disegno di legge nel suo complesso. Le Commissioni torneranno a riunirsi nelle giornate del 7 e 8 gennaio 2021, senza limitazioni di materie collegate all'emergenza epidemiologica. L'Assemblea tornerà a riunirsi martedì 12 gennaio 2021, alle ore 16,30, con ratifiche di accordi internazionali definite in Commissione. Capigruppo è convocata nello stesso giorno dalle ore 15.

a far sapere che da parte del Gruppo Lega non c'è stata alcuna particolare opposizione nella stesura del calendario appena letto. Allo stesso tempo, però, prendiamo atto con rammarico che per la prima volta nella storia della Repubblica una manovra economica arriva qui al Senato in seconda lettura il 27 dicembre. Questo è davvero drammatico per la democrazia del nostro Paese, perché non ci sarà assolutamente la possibilità

volta il Presidente del Senato - lei - annuncia l'assegnazione del disegno di legge, della manovra di bilancio alla Commissione

per evitare l'esercizio provvisorio, questa volta abbiamo dimostrato con i fatti il vero senso di responsabilità che abbiamo nei confronti del Paese e delle tante categorie che in questo momento stanno soffrendo. Lo facciamo per loro, perché voi

il decreto-legge in esame, composto da due capi e da dieci articoli, detta misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della Regione Calabria (capo I) e per il rinnovo degli organi elettivi delle Regioni a statuto ordinario (capo Il capo I, che va dall'articolo 1 all'articolo 7, interviene a sostegno della gestione del sistema sanitario della Regione Calabria allo scadere, lo scorso 3 novembre, dell'efficacia delle disposizioni del decreto-legge n. 35 del 2019, prevista in diciotto mesi dalla sua entrata in vigore (3 maggio 2019). L'intervento è disposto considerata la perdurante criticità del sistema sanitario calabrese determinata dal mancato raggiungimento dell'equilibrio Le norme in esame, di cui al capo I, si applicano fino all'11 novembre 2022 ovvero, come specificato dalla Camera, fino ad un termine anteriore a tale data, in caso di raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, Questi ultimi sono gli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale. L'articolo 1 stabilisce le funzioni del commissario *ad acta* nominato dal Governo, chiamato ad attuare gli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della Calabria a svolgere, ove delegato, i compiti di rafforzamento strutturale della rete ospedaliera del servizio sanitario, con l'adozione di specifici piani di riorganizzazione per far fronte all'emergenza Covid e assicurare l'attuazione delle misure del decreto in esame. Il commissario *ad acta* è coadiuvato, ai sensi del successivo comma 3, da uno o più subcommissari, il cui numero non può essere superiore a Il comma 2 dello stesso articolo 1 concerne le dotazioni di personale, di uffici e di mezzi che la Regione Calabria è tenuta a mettere a disposizione del commissario *ad acta*. Il comma 4 prevede che il medesimo commissario si avvalga del supporto tecnico e operativo dell'Agenzia attraverso personale comandato, nel limite di 12 unità, o attraverso contratti di lavoro flessibile, nel limite di 25 unità. In caso di inadempienza della Regione nel fornire il necessario supporto, il commissario *ad acta*, dopo averne dato comunicazione al Consiglio dei ministri, invita la Regione a svolgere i suoi compiti entro il termine previsto (massimo in trenta giorni) e, se perdura l'inadempienza, è prevista l'attivazione dei poteri sostitutivi dello Stato. Il successivo comma 4-*bis* prevede che al fine di garantire l'esigibilità dei livelli essenziali di assistenza nella Regione Calabria, il Ministro della salute, al verificarsi delle condizioni di cui al successivo articolo 6, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del Servizio sanitario regionale e sentito il commissario *ad acta*, autorizzi quest'ultimo ad un piano straordinario per l'assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza, facendo ricorso innanzitutto agli idonei delle graduatorie in vigore, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente relativi agli oneri per il personale del Servizio sanitario nazionale e nel rispetto del limite di spesa di 12 milioni annui a decorrere dal 2021. L'articolo 2 prevede la nomina di commissari straordinari per ogni ente del Servizio sanitario della Calabria. Alla nomina provvede il commissario *ad acta* previa intesa con la Regione, nonché con il rettore nei casi di aziende ospedaliero-universitarie. Il comma 4 del medesimo articolo 2 prevede che entro novanta giorni dalla nomina, i commissari straordinari adottino l'atto aziendale avente ad oggetto la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'azienda, che è successivamente approvato dal commissario *ad acta*, ed approvino i bilanci aziendali relativi agli esercizi già conclusi. Il comma 5 definisce le procedure sostitutive per i casi di mancato rispetto del suddetto termine a cui conseguono in ogni caso, ai sensi del comma 6, la decadenza automatica dall'incarico e l'esclusione del riconoscimento del compenso aggiuntivo. Il comma 7 concerne le procedure di sostituzione dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario della regione Calabria. Il comma 8 prevede informative periodiche da parte di ciascuno dei commissari straordinari alla Conferenza dei sindaci e alle organizzazioni sindacali. L'articolo 3 disciplina le procedure per l'affidamento di appalti, lavori e forniture per gli enti del Servizio sanitario regionale della Calabria e il programma operativo per la gestione dell'emergenza Covid e per l'edilizia sanitaria. In particolare, il comma 1 disciplina le procedure per l'affidamento di appalti, lavori e forniture per gli enti del Servizio sanitario regionale; il comma 2 pone un termine per la predisposizione sia del programma operativo per la gestione dell'emergenza Covid sia del Piano triennale straordinario per l'edilizia sanitaria e l'adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale; il comma 3 disciplina l'attuazione dei progetti di edilizia sanitaria. A tal fine, il commissario *ad acta* si avvale degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla società Consip. Inoltre, il commissario *ad acta* può delegare l'espletamento delle procedure in questione ai suddetti commissari straordinari. Il comma 2 prevede che il commissario *ad acta* adotti, nel termine di trenta giorni dalla sua nomina, il programma operativo per la gestione dell'emergenza Covid e definisca, nel termine di sessanta giorni dalla nomina, il piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale regionale. Come previsto dal comma 3, gli interventi in materia di edilizia sanitaria, finanziati da risorse statali, sono attuati dal commissario straordinario. L'articolo 4 concerne l'eventuale scioglimento di singoli enti del Servizio sanitario della Calabria ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il cosiddetto TUEL. In particolare, il comma 1 prevede che nel caso di adozione dei provvedimenti di scioglimento summenzionati, la commissione straordinaria per la gestione dell'ente, nominata con decreto di scioglimento dell'ente medesimo, operi a garanzia dei livelli essenziali di assistenza, in coordinamento con il summenzionato commissario *ad acta*, nonché in conformità con gli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo

per le questioni tecnico-sanitarie, di un soggetto di comprovata professionalità ed esperienza in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, nominato dal Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro della salute. Ai sensi del comma 3, la commissione straordinaria può avvalersi in via temporanea, in posizione di comando o di distacco, di esperti nel settore pubblico sanitario nominati dal prefetto, su proposta del Ministro della salute. Il comma 4, sempre per le ipotesi di aziende sanitarie sciolte, demanda alla suddetta commissione straordinaria per la gestione dell'ente l'adozione dell'atto aziendale e l'approvazione dei bilanci aziendali relativi agli esercizi già conclusi. Il comma 1 e il comma 1-*bis* dell'articolo 5 concernono rispettivamente la collaborazione del Corpo della guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate con il commissario *ad acta*. Il comma 1 dell'articolo 6 prevede che, al fine di supportare gli interventi di potenziamento del servizio sanitario della Calabria, sia accantonata, a valere sulle risorse nazionali destinate all'attuazione dei progetti di carattere prioritario in ambito sanitario, una somma di 60 milioni di euro a favore della Regione stessa per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il comma 2 dell'articolo 7 prevede che il commissario *ad acta* invii al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze ogni sei mesi una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente capo 1, anche con riferimento all'attività svolta dai commissari straordinari. Il capo 2 (articoli 8-10), infine, detta disposizioni urgenti per il rinnovo degli organi elettivi delle Regioni a statuto ordinario. L'articolo 8 detta disposizioni sui termini entro i quali hanno luogo le consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi. In particolare, il comma 1 dispone che le elezioni degli organi elettivi si svolgano non prima del novantesimo giorno e non oltre il centocinquantesimo successivo alla data in cui si siano verificate le circostanze che rendono necessario il rinnovo ovvero nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.

Signor Presidente, Governo, cari colleghi e colleghe, questo provvedimento è il passo seguente al primo decreto Calabria del nostro ministro della salute Grillo per rilanciare il servizio sanitario della Regione.

mettere il *focus* su questa situazione non è soltanto necessario, ma assolutamente doveroso per Governo e Parlamento. È un momento delicatissimo per il Paese: l'emergenza Covid ha messo a nudo con violenza tutte le fragilità del nostro Sistema sanitario nazionale. Quindi non possiamo più perdere tempo; bisogna intervenire con misure straordinarie, concrete e risolutive. Il decreto-legge oggi in discussione al Senato va in questa direzione; sia le ragioni che gli obiettivi sono assolutamente condivisibili. Ritengo pertanto che questo decreto-legge vada oltre la Calabria e rappresenti anche un gesto di grande attenzione per tutto il Sud Italia. Io vengo dalla Sicilia, precisamente da Sciacca, dove ho esercitato la professione medica anni, precisamente nel pronto soccorso dell'ospedale della mia città. Conosco quindi molto bene tutte le disfunzioni e le criticità, perché le ho vissute sul campo e le ho condivise ogni giorno e ogni minuto con i pazienti, che troppo spesso, nonostante i nostri grandi sforzi come personale medico, si sono trovati di fronte a situazioni inaccettabili, causate da evidenti falle del nostro sistema sanitario. Noi tutti siamo impegnati per dare una migliore sanità al nostro Paese e ai cittadini italiani. In questi mesi infatti abbiamo approvato un notevole numero di decreti di importanza straordinaria per il settore sanitario, con due obiettivi di fondo: ridare centralità al Servizio sanitario pubblico con una serie di ingenti investimenti e caratterizzare l'assistenza socio-sanitaria con un principio di fondo, ovvero la territorialità. Questo considerevole impegno istituzionale è iniziato ben prima dell'arrivo dell'emergenza Covid, segno evidente di quanto la sanità italiana avesse bisogno di una profonda riforma, all'insegna dell'innovazione e del maggiore ascolto dei principali bisogni del cittadino. Da troppe parti, infatti, si levava forte la necessità di radicali trasformazioni, a partire dai nostri ospedali pubblici, ormai non più sufficienti ad assecondare tutti i bisogni sanitari, passando per il personale medico e infermieristico, in cronica carenza di risorse umane, per finire con gli inadeguati supporti tecnologici, fermi da decenni. Il nostro Servizio sanitario nazionale, enorme e storica ricchezza del nostro Paese, ha subito così un certo rallentamento negli ultimi anni. anni. Era quindi assolutamente necessario ed indispensabile - e lo è ancora - uno scatto in avanti, a cominciare proprio da qui, dal cuore delle istituzioni, ovvero da quel luogo dove devono essere concepite ed approvate le riforme legislative, che possano consentire ai servizi territoriali di uniformarsi verso livelli più adeguati ai reali bisogni sanitari della cittadinanza. È quello che da tempo stiamo facendo, anche con il decreto-legge oggi al nostro esame, a cui vai il nostro pieno e convinto appoggio. Certamente questo vento di riforme in campo sanitario dovrà continuare, se possibile, con ancora più forte condivisione. Tra le misure da evidenziare c'è la previsione che il Ministero della salute possa autorizzare il commissario *ad acta* ad adottare un piano di assunzioni straordinario di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore dell'emergenza e urgenza, facendo ricorso innanzitutto agli idonei delle graduatorie in vigore, con una spesa di 12 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021. Sappiamo che negli ultimi dieci anni sono stati fatti tagli alla sanità per 37 miliardi di euro. Sappiamo che il MoVimento 5 Stelle, da quando è arrivato al Governo, ha invertito questa rotta, sappiamo che nell'ultimo anno abbiamo stanziato quasi 12 miliardi di euro, ma sappiamo anche che la sanità,

ovvero il Governo, il Parlamento, le stesse Regioni, gli enti territoriali e locali e le parti sociali. Sarà quindi necessaria una concertazione vasta e diffusa, affinché si arrivi a un modello di Servizio sanitario veramente a misura di cittadino e delle sue fragilità. Questo sarà il vero salto di qualità da compere, evitando la frammentazione dei servizi e il disorientamento dei pazienti, puntando invece ad una ottimizzazione delle risorse economiche. Per fare questo, *in primis*, si dovrà ridurre l'ospedalizzazione, laddove non necessaria, puntando altresì ad una ricerca scientifica, che possa usufruire di finanziamenti più importanti e ad una prevenzione sanitaria che possa svilupparsi attraverso strumenti sempre più avanzati e moderni. E ancora, si dovrà puntare ad un'assistenza al paziente, che inizi dalla sua abitazione, ovvero dal luogo più caro e confortevole, in un percorso completo, che possa svilupparsi partendo dal medico di base, evitando così inutili trasferimenti in ospedale, che sottopongono il paziente e i familiari ad uno *stress*, che sicuramente comporta negative ripercussioni a livello psicofisico. Questa fondamentale esigenza è stata pienamente raccolta in questa legislatura, con importanti misure nel segno della concretezza e dell'ascolto dei bisogni della collettività. Ad esempio, nel decreto-legge rilancio, il Governo ha previsto l'assunzione di 9.600 infermieri, istituendo la figura dell'infermiere di famiglia, ma non tutte le Regioni hanno provveduto a queste assunzioni. Non parlo degli infermieri di famiglia a caso, perché proprio per istituire questa figura ho ritenuto quanto mai utile e opportuno presentare uno specifico disegno di legge. Adesso che il Governo è intervenuto, è necessario però che questi infermieri entrino davvero a far parte dei Servizi sanitari territoriali, su cui noi del MoVimento 5 Stelle insistiamo da anni. La sanità del futuro si dovrà basare sulla medicina territoriale, per alleggerire gli ospedali e fare in modo che ci si rivolga ai nosocomi solo per le emergenze e le malattie, che davvero necessitano di un ricovero. Questa è la grande sfida che ci aspetta e che siamo pronti a raccogliere.

decreto Calabria-*bis* rappresenta la palese sconfitta delle politiche commissariali attuate negli ultimi anni e la decisione del Governo di adottare l'ennesimo decreto-legge si pone, a mio avviso, in palese contrasto con i principi costituzionali più volte ribaditi dalla Consulta. Quest'ultima, nel pronunciarsi, con la sentenza n. sulla costituzionalità relativa al primo decreto Calabria, ha affermato che il provvedimento normativo d'urgenza costituiva un intervento normativo non ordinario, ma appunto straordinario, che si proponeva di affrontare con determinazione e rapidità il tentativo di traghettare la sanità calabrese verso la normalità, dotando il commissario *ad acta* di poteri per l'attuazione degli obiettivi del Piano di rientro e soprattutto per rimuovere la sistematica violazione degli obblighi derivanti dai principi della funzione pubblica, gestione del personale fuori controllo e le diverse divergenze tra vertici politici regionali e struttura commissariale, con il risultato di una griglia dei LEA peggiore di ogni altra Regione. presupposti non sarebbero serviti a nominare un nuovo commissario, atteso che la Regione Calabria, a seguito delle elezioni del 2020, ha intrapreso un percorso virtuoso, volto a ricondurre la gestione del servizio sanitario regionale a canoni di efficienza ed efficacia. Per questo motivo, l'emanazione di un nuovo decreto-legge ha leso gravemente le competenze regionali in termini di salute, le quali vengono violate non solo temporaneamente ed eccezionalmente contratte in ragione della pregressa inerzia regionale o comunque del non adeguato esercizio di competenze, come affermato dalla sentenza della Corte costituzionale. Nelle ultime settimane abbiamo assistito a un teatrino inverosimile connesso alle nomine di un commissario. c'era già un professionista, voluto dalla presidente Jole Santelli, alla quale rivolgo un pensiero commosso, perché oggi compirebbe Assistiamo comunque al fallimento del precedente provvedimento, che ha visto l'incapacità della gestione commissariale di raggiungere i risultati attesi. È aumentato il debito e sono peggiorati ulteriormente i LEA. Alla fine è arrivato il prefetto Guido Longo e speriamo che si possa finalmente vedere un epilogo positivo di questa grottesca vicenda, che ancora una volta ha dimostrato l'incapacità e la sprovvedutezza del Governo che ha deciso tutto questo. La gestione commissariale della sanità calabrese va avanti da dieci anni, durante i quali è peggiorata la qualità dei servizi erogati, sono aumentati i viaggi della speranza dei calabresi (ossia la mobilità passiva) e si sono progressivamente visti uno svuotamento e un abbandono degli ospedali e la mancanza di figure importanti come medici e infermieri a causa del blocco del *turn over*.

che, a fronte dei tanti sacrifici finanziari, non godono di servizi adeguati. Nella relazione la magistratura contabile ricorda di avere da anni rimarcato le patologie della sanità calabrese, che, come dicevamo, non ha approvato i bilanci. Gli ultimi atti ufficiali del bilancio risalgono al 2014. Dieci anni dopo l'adozione del Piano di rientro - cioè a fine 2019 - il disavanzo sanitario è passato a circa 225 milioni di euro. La magistratura contabile ricorda che il punteggio dei LEA tradisce ancora numerose anomalie evidenzia che il disavanzo sanitario, a differenza di quello accumulato da un Comune, non mette in pericolo i livelli dei servizi pubblici di un territorio, ma pregiudica la realizzazione dei livelli essenziali di assistenza per tutti gli abitanti di una Regione, mettendo in pericolo la tutela del diritto alla salute dei calabresi. Alla luce di questa relazione impietosa, mi chiedo quale sia stata la *ratio* che ha portato non solo a rinnovare il commissariamento, ma addirittura ad aumentarne i termini a ventiquattro mesi. Bisognava avere fiducia e scommettere sul Governo regionale e sui cittadini, ma, forse, essendo un Governo di centrodestra - che vincerà nuovamente le prossime elezioni nazionale vuole accentrare tutto il potere e le poltrone disponibili. E pensare che il 13 settembre il presidente Jole Santelli aveva inviato una lettera accorata

il rispetto dei LEA e il rispetto di obiettivi economico-finanziari, ma è necessaria una *governance* con competenze manageriali specifiche per la materia sanitaria, con una visione che non si acquisisce soltanto con una poltrona occupata, ma con una formazione specialistica. A questo punto, non resta che rimarcare tre priorità che dovranno essere perseguite: la prima, coinvolgere tutti i livelli istituzionali (Stato, Regioni e aziende) e superare le conflittualità; la seconda, a fronte dell'assunzione straordinaria di personale, costruire una forte motivazione e un'identità aziendale, orientata agli obiettivi che devono essere comunicati e verificati periodicamente (naturalmente, tutti gli emendamenti a questo proposito che abbiamo presentato in Commissione sanità, anche oggi, sono stati respinti); la terza, verificare i fabbisogni, a cui si deve affiancare un sistema di misurazione della *performance*, con pochi indicatori attendibili e coerenti. Vorrei sottolineare che la Calabria è soltanto la punta di un iceberg nel panorama sanitario del nostro Paese e, alla luce dell'esperienza vissuta e che viviamo della pandemia, che la tutela della salute è legata anche alla tutela dell'economia e del benessere di un Paese: altro che redditi di cittadinanza ai mafiosi! E mi permetto di ribadire che i 9 miliardi destinati dal *recovery fund* alla sanità sono una cosa ridicola, meno che il Governo non abbia già deciso - bene! - di prendere i 37 miliardi del MES. Per concludere, vorrei evidenziare due aspetti inaccettabili che sono stati volutamente fatti passare inosservati: il primo riguarda il potere che il commissario Arcuri ancora una volta avrà nel gestire fondi pubblici senza essere controllato e senza poter essere accusato di alcunché grazie allo scudo legale che l'emergenza sanitaria gli ha concesso. trovo scandaloso che il Governo continui ad affidare al commissario Arcuri deleghe in bianco praticamente su tutto lo scibile umano *(Applausi)*, senza avere di ritorno un adeguato modello di efficienza, trasparenza e tempestività. In questo decreto-legge vengono affidati ad Arcuri - e, per suo tramite, a Invitalia - 440 milioni di euro per l'edilizia sanitaria e l'ammodernamento tecnologico. Come noto, il commissario, in considerazione del suo ruolo, gode dello scudo penale, quello scudo che finora è stato negato a medici e personale sanitario in trincea fin dai primi giorni di questa pandemia e anche adesso oggetto di numerosi attacchi negli ospedali da parte dei cittadini esasperati. Questo vorrà dire che Arcuri potrà disporre di risorse enormi senza che i calabresi per primi sappiano perché cosa verranno usate. anche le ultime vicende perché Arcuri è comunque il commissario delle mascherine sbagliate, delle mascherine fantasma, delle gare d'appalto per i banchi a rotelle (arrivati a scuole chiuse), di cui da mesi chiediamo, con interrogazioni parlamentari, di avere l'onore di conoscere il prezzo

con la promessa che dopo dieci anni di precariato avrebbero visto la loro professionalità premiata. È tuttora assordante il silenzio delle istituzioni di fronte a queste settanta famiglie di lavoratori che fra tre giorni saranno a casa. Avete stabilizzato chiunque, ma questi settanta lavoratori vi danno fastidio *(Applausi)*, perché sono professionalità che lavorano nell'Agenas e che danno fastidio a chi vuole soltanto avere dei passacarte. Un'amministrazione che è stata svilita ed esautorata dalle sue funzioni per almeno sei mesi in piena emergenza sanitaria e che continua ad essere mortificata con la perdita di settanta precari con un *know-how* scientifico e tecnico decennale.

un dirigente ogni sette dipendenti. Mi sembra un po' troppo per chiunque. Il Governo con il disegno di legge di bilancio non ha dato seguito alle rassicurazioni che avevano avuto questi settanta lavoratori, ma credo che anche qui andrà avanti la procura della Repubblica, in quanto il commissario attuale verrà denunciato dai precari dell'Agenas. *(Applausi)*.

è sottoposta, purtroppo da oltre dieci anni, al piano di rientro sanitario. Tanti cittadini non riescono ad usufruire del diritto costituzionale alla cura e sono costretti alla migrazione sanitaria, che comporta pure un incremento di spesa e quindi un rischio di sforamento di *budget*. Purtroppo, ben 300 milioni all'anno all'anno del *budget* sanitario calabrese vanno a finire in altre Regioni per sopperire alle carenze nella garanzia di un sistema sanitario efficiente della Regione Calabria; sistema sanitario che purtroppo è estremamente carente. Si sono avvicendati diversi commissari governativi per gestire la situazione, gravemente compromessa da troppi anni di malagestione. Non a caso ci ritroviamo ben due ASP commissariate per infiltrazioni mafiose, quella di Reggio Calabria e quella di Catanzaro. Non tutti sapranno o ricorderanno che i bilanci di quattro anni dell'ASP di Reggio Calabria sono spariti e sono stati sostituiti da bilanci orali. Non tutti forse sapranno che il commissariamento governativo ha riguardato solo l'aspetto economico-finanziario, ma quello gestionale è sempre rimasto nelle mani della Regione Calabria, ed i Governatori che si sono susseguiti hanno sempre confermato le stesse persone alla guida delle ASP, così come hanno sempre confermato premialità per tutti i dirigenti che, dopo numerosi anni di questa gestione, hanno portato l'indice dei LEA a 136, ovvero ben 24 punti al di sotto delle soglie di accettabilità. Quali sono le principali cause del dissesto? Bisogna risalire alle cause, e non giudicare gli effetti ed attribuire la responsabilità a chi oggi sta cercando di porre rimedio. Il rapporto malato pubblico-privato, per il quale si faceva ricorso a continui sforamenti del *budget* destinato a strutture private convenzionate con la compiacenza dei dirigenti sanitari e con conseguente contenzioso e nuovi oneri per il bilancio delle ASP; le forniture spesso inutili ed obsolete, pagate fuori da listini di mercato e liquidate anche più volte; assunzioni clientelari da parte dei politici di turno: tutto ciò ha subito una inevitabile battuta d'arresto con il commissariamento governativo, ma ha anche comportato delle restrizioni non indifferenti sul diritto alla cura dei calabresi, che si sono visti improvvisamente aumentare il costo delle prestazioni della diagnostica ed imporre limitazioni nelle prescrizioni (questo è stato un effetto, purtroppo). Oggi per la seconda volta votiamo un decreto per la sanità calabrese. Abbiamo reso la struttura commissariale più incisiva anche nel merito della gestione del servizio sanitario grazie a un suo potenziamento sotto il profilo amministrativo e sanitario. Le precedenti strutture commissariali hanno sempre operato in una sorta di deserto istituzionale e in contrasto con il Governatore di turno,

Adesso il commissario sarà supportato da una struttura fino a tre commissari, altri subcommissari, da un contingente minimo messo a disposizione dalla Regione Calabria di altri 25 elementi, più il supporto del personale dell'Agenas. È stata data disponibilità a effettuare un piano assunzionale sanitario e socio-sanitario straordinario per cui è stato stanziato un *budget* di 12 milioni di euro all'anno a partire dal 2021 da destinarsi alla nostra Regione. Inoltre, per il piano di rientro sono stati stanziati altri 180 milioni per i debiti certificati, ma non so quanti sono quelli non certificati a causa dei bilanci mancanti e speriamo che il commissario adesso venga a capo di questo groviglio inestricabile. Tutto ciò indica quanto sia necessaria la vigilanza dello Stato sui sistemi sanitari regionali e quanto è indispensabile che le dirigenze sanitarie vengano assunte non dalla politica, ma in base a concorso pubblico e a criteri meritocratici e non di affiliazione politica. fondamentale rivedere i parametri di assegnazione dei fondi per il finanziamento dei servizi sanitari regionali sulla base non della popolazione pesata, ma anche in funzione delle comorbilità, che sicuramente comportano costi di gestione più elevati. È fondamentale che il Sistema sanitario nazionale possa essere sostenuto attraverso l'impiego di strutture pubbliche a copertura di tutto il fabbisogno. Le strutture private che hanno gestito male le risorse e che rischiano la chiusura perché hanno operato gonfiando le spese a carico del servizio sanitario regionale, se attualmente indispensabili a garantire la continuità del servizio dell'assistenza per alcune prestazioni sanitarie, devono essere pubblicizzate. Questa è la ricetta per uscire dalla drammatica situazione in cui oggi si trova non solo la sanità calabrese, ma la sanità di tante altre Regioni italiane.

andrò controcorrente dai banchi della maggioranza impegnando solo me stesso nelle cose che dirò sul decreto Calabria. Mai come ora sento l'orgoglio e la responsabilità di essere sindaco e, al contempo, come senatore della Repubblica calabrese, non posso che sentirmi mortificato e deluso da un Governo che, di fatto, sembra aver dimenticato e abbandonato la Calabria, la Calabria, che è sempre più considerata la Cenerentola d'Italia. Ancora una volta, l'Istat ci racconta di un Sud e di una Calabria spogli di servizi in cui gli ultimi continuano a restare ai margini, immersi in una lotta per la sopravvivenza, dove i diritti primari, come quelli al lavoro, alla salute all'istruzione, non riescono a trovare piena realizzazione. Sono solo uno tra i tanti sindaci calabresi che quotidianamente indossano la fascia tricolore con quella passione e quella determinazione indispensabili per affrontare il difficile percorso amministrativo e che in trincea, giorno e notte, si impegnano al massimo senza le risorse necessarie cui hanno diritto, ma con tutta la forza e l'energia che possiedono, facendo il possibile e anche l'impossibile per i propri cittadini che vedono in loro l'unico, vero e fondamentale punto di riferimento a cui aggrapparsi e rivolgersi per ogni esigenza, specialmente in questo periodo. Oggi più di ieri noi sindaci siamo alle prese con la difficoltà di far quadrare il difficile equilibrio tra domanda dei cittadini e offerta pubblica. Ci misuriamo con piccoli e grandi problemi della nostra gente, ascoltiamo la loro disperazione, cerchiamo di rielaborarla in soluzioni e, soprattutto, non ci voltiamo mai dall'altra parte. Siamo sempre noi ad accogliere le ansie di ogni madre, le preoccupazioni di ogni padre, le inquietudini di ogni ragazzo, le aspirazioni e i progetti di vita di ogni giovane e a raccogliere il grido di aiuto di uomini, donne, anziani, giovani e, purtroppo, bambini, costretti a lasciare la Calabria ed affrontare l'esodo sanitario verso gli ospedali del Centro-Nord, un calvario personale e familiare, per farsi curare da malattie oncologiche, sottoporsi a visite specialistiche e operazioni chirurgiche. Era questo il senso ed il motivo del mio emendamento al cosiddetto decreto Calabria, in cui proponevo di istituire all'interno della struttura commissariale sulla sanità un organo formato da sindaci, con poteri di controllo e di proposta. Allo stato dei fatti però tale emendamento - non solo mio perché ha la voce, il volto e l'anima di tantissimi sindaci calabresi - è stato stravolto totalmente e privato della parte in cui si prevedeva un diretto coinvolgimento dei sindaci nella filiera di comando della struttura commissariale della sanità. Mi sono a lungo speso perché tale previsione venisse inserita nella parte normativa, convinto che le amministrazioni locali siano le sole a conoscere i reali servizi sanitari sui territori e, quindi, in grado di contribuire a una concreta risoluzione delle tante questioni aperte nella sanità calabrese. Purtroppo questa norma è stata inopinatamente stralciata e ciò dovrebbe preoccupare l'intera delegazione dei senatori calabresi, quantomeno di coloro che appartengono al centrosinistra e alla maggioranza di Governo. Sono questi i temi in cui si misura la qualità dei gruppi dirigenti, di chi nutre l'ambizione di governare la Calabria e di chi ha veramente a cuore il destino della Regione.

soprattutto guardando al dibattito che sta prendendo piede in Calabria in vista delle elezioni regionali, con un confronto completamente sganciato dalla realtà, privo di contenuti e finalizzato solo all'autoconservazione. Il passato ci insegna che una classe politica conservatrice, preoccupata di difendere lo *status quo,* è capace solo di scrivere le pagine più brutte della nostra storia regionale e nazionale. Il futuro ci sollecita a lanciare un segnale di grande maturità e coerenza, dando dimostrazione di avere nel cuore e nella mente solo ed esclusivamente il bene e la crescita della nostra Nazione, di cui fa parte anche la Calabria, una terra dalla storia millenaria, che coincide con quella dell'umanità, dove si respira l'anima di una civiltà che vive in una cultura che è storia, Magna Grecia, Italia. Una Regione che è già in ginocchio economicamente e socialmente di suo, rischia così di ricevere il colpo finale con un decreto vacuo e vuoto che non riesce a garantire il diritto costituzionale alla salute, ai livelli di assistenza, di prevenzione e di cura pari alle altre Regioni, a colmare il profondo divario tra Sud e Nord, a ripianare i debiti esistenti, a contemplare risorse per investimenti in capitale umano e tecnologia. Pertanto, proprio per tutelare fino in fondo i diritti dei calabresi, sono mio malgrado costretto a votare no al cosiddetto decreto Calabria. Se votassi il testo del decreto, così come è stato modificato nei lavori parlamentari alla Camera, tradirei me stesso, la mia gente, le mie radici, la mia storia, i miei ideali: quegli ideali che ho scelto di servire da quando avevo quattordici anni, mettendoci non solo la faccia, ma anche il cuore e agendo per il bene nell'esclusivo interesse della collettività. nostro esame doveva rappresentare una svolta per la sanità in Calabria; in realtà si tratta di una norma anemica, che non cura i mali prodotti dalla gestione nefasta dei governi regionali prima e, a partire dal 2010, del commissariamento calabrese, di un'amministrazione inconcludente, parolaia, superficiale e senza bussola dello Stato italiano. Il decreto-legge doveva esaltare il ruolo dei sindaci, e invece li umilia, mandandoli contemporaneamente in prima linea a mani nude. In più l'attuale pandemia ha aumentato a dismisura il peso di chi ha l'onore e l'onere di indossare la fascia tricolore, riservata non ai parlamentari, non ai Ministri, non al Presidente del Consiglio, ma solo ai primi cittadini delle nostre martoriate comunità. In questo decreto-legge non viene valorizzata la funzione fondamentale dei rappresentanti veri e autentici del territorio, come avevo chiesto a gran voce in rappresentanza di tutti i sindaci calabresi. Anzi, viene tolto anche quello che il decreto legislativo n. 502 del 1992 e le successive modifiche avevano previsto. Un esempio per tutti: viene di fatto svuotato il parere preventivo nella nomina dei direttori generali che la Conferenza dei sindaci doveva esprimere. Il decreto-legge non prevede in maniera puntuale e precisa i requisiti specifici, attinenti al settore, che deve possedere il commissario regionale; non individua i titoli che devono avere i componenti della sua catena di comando; si muove sulla linea sottile dell'incostituzionalità, perché incide profondamente sui delicati equilibri che tengono insieme lo Stato e il regionalismo. Quello in esame è un decreto-legge che rappresenta uno sfondamento dei poteri istituzionali in capo al rappresentante della collettività calabrese, cioè al Presidente della Regione; uno sfondamento costituzionale che proviene da chi si è battuto senza ragione contro la riforma costituzionale, in virtù dei presunti valori che prima difendeva legittimamente e oggi vuole tradire in maniera strisciante e silenziosa. È vero che la situazione sanitaria è emergenziale in Calabria; lo Stato però da più di dieci anni governa e amministra tale realtà e non può immaginare di scaricare sulla Calabria, sia politicamente, ma soprattutto economicamente, i disastri finanziari. in esame c'è in verità un tentativo di intervento economico, ma è timido e insufficiente. Lo Stato deve addossarsi tutto e per intero il disavanzo degli ultimi dieci anni, perché è il frutto della gestione dello Stato stesso, attraverso i suoi commissari. *(Applausi)*. Con il provvedimento in discussione si vuole governare per sempre la Calabria attraverso la sanità; di fatto, si stabilisce un principio che anche la moderna civiltà giuridica avanzata aborre: il fine pena mai. il fine commissariamento in Calabria mai. Sono cresciuto alla scuola di quella politica, che parte dal basso ed è fatta con dignità, coerenza e trasparenza, in una piccola sezione del Partito Socialista, in piazza, per la gente e tra la gente. Per È questo il modo di essere e di fare politica a cui ho sempre creduto, ispirandomi a una donna tenace e coraggiosa, un grande esempio di passione e disinteressato impegno civile, culturale e sociale per la sua terra in difesa dei diritti dei cittadini, in particolare delle fasce più deboli delle popolazioni: l'unica donna

Allora quella donna ci è riuscita, a differenza di oggi, quando il diritto alla salute viene garantito con tagli e chiusure di strutture ospedaliere, che paradossalmente peggiorano l'efficienza sanitaria e aumentano il *deficit* pubblico. Quella straordinaria donna è una calabrese, Marianna Presta, mia madre, interprete autentica dei veri valori e dei più alti ideali della tradizione socialista *(Applausi)*, che incarna nella propria storia la politica autentica, quella che mette al centro la persona e l'amore per la *polis*; la politica in cui mi riconosco e a cui sono fiero di appartenere, con cui ho sempre operato e con cui sto svolgendo la mia attività di parlamentare e con cui amministro da sindaco. Tuttavia, se, come sembrerebbe, la politica sta diventando tutt'altra cosa, con l'amarezza di chi ha creduto e crede nel valore delle istituzioni, con la responsabilità civile e morale che appartiene alla mia cultura e coerenza politica di cittadino, di uomo libero e democratico, valuterò il mio ritiro dall'attività politica al termine della legislatura parlamentare e del mio mandato da sindaco. Mi sentirei decisamente a disagio all'interno di un così machiavellico e arido contenitore della politica. Buone feste a tutti quanti. *(Applausi)*. PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bini. Ne ha facoltà. Signor Presidente, sarò molto più breve dei colleghi che mi hanno preceduto, perché poi ci sarà tempo anche in occasione delle dichiarazioni di voto finale

- il che di per sé mi pare significhi che neanche chi l'aveva presentata probabilmente fosse molto convinto della bontà degli elementi di incostituzionalità presenti comunque ci ha ricordato, in occasione dell'ultimo decreto-legge, che, quando ci sono problemi legati ai servizi essenziali ai cittadini, è normale che lo Stato debba intervenire. È proprio la nostra Costituzione che garantisce questo elemento e che, rispetto a un tema di materia concorrente, quando però non si riescono a garantire quei servizi essenziali e soprattutto che siano pari

possa avere la stessa qualità delle cure. Ad oggi non è così: ce lo dobbiamo dire. Lo vediamo tutti, e non solo in Calabria, dove però vi è una situazione particolare, relativa non solo a un elemento di conti

ma c'è anche un elemento, che non si può sottacere in quest'Aula, che vede una connessione non positiva tra il mondo politico, quello della sanità calabrese e infiltrazioni malavitose. Lo abbiamo visto più volte, in questi anni, ricorrere anche nelle cronache nazionali. È un elemento che, secondo me, deve spingere e portare al commissariamento esterno. Più ci sono elementi di natura, di concomitanza e di relazioni strane nel territorio, più è importante che venga qualcuno che ha una terzietà per poter gestire

e anni nei quali ricordo che, almeno gli ultimi due decreti, sono stati approvati da due maggioranze diverse. Probabilmente, anche questo dovrebbe far riflettere sul fatto che, più che dedicarsi a una polemica politica o alla necessità, da calabresi (non essendolo, sono più libera, da questo punto di vista), di far vedere al territorio che si difendono gli interessi del pezzettino di paese che si rappresenta, si dovrebbe avere, forse, la capacità di rendersi conto che c'è da fare uno scatto in più. C'è bisogno di restituire dignità ai cittadini calabresi che non hanno un colore politico. Non bisogna farne una questione politica, ma bisognerebbe provare tutti - con la dovuta collaborazione istituzionale, in cui il Governo deve fare la propria parte in relazione con gli altri enti e le altre istituzioni - a restituire alla Calabria la sanità che merita. Questo è l'elemento fondamentale per cui ci sentiamo di sostenere questo decreto-legge. la Calabria non è una terra banale. Solo se si tiene bene a mente questa valutazione sarà possibile, anche sul tema che stiamo discutendo e affrontando oggi, giungere a idee e proposte per superare la crisi. Nei giorni che hanno preceduto questo dibattito si è sentito di tutto e il contrario di tutto. Non vi è dubbio che la sanità in Calabria abbia avuto una vicenda travagliata, perché le contraddizioni, le difficoltà economiche, il tessuto sociale disgregato, la fragilità della produzione, anche i condizionamenti della criminalità organizzata e i lacci e lacciuoli del passato hanno un peso specifico assolutamente negativo sul presente. Tutto ciò, com'è stato ricordato, ha portato a dieci anni di commissariamento, con risultati tutt'altro che edificanti. L'approccio dei commissari - mandati dal Governo e non dalla gente calabrese - è stato, nella migliore delle ipotesi, ragionieristico

Questi tagli si sono tradotti in un vero e proprio *vulnus*, di cui è responsabile la politica, e in un depauperamento dell'offerta sanitaria, che merita la più ampia e profonda censura. È anche vero che il debito della sanità, prima del commissariamento, aveva raggiunto livelli di guardia non più sostenibili, ma l'intervento dello Stato, quello che ancora oggi auspicate, non ha fatto che aggravare la situazione in Calabria, perché nella logica del commissariamento c'è qualcosa che non quadra ed è proprio l'approccio. Da un lato, si operano tagli su tagli, che condannano i pazienti calabresi a una sempre crescente migrazione sanitaria, e dall'altro, in caso di necessità, il sistema sanitario calabrese ha dimostrato debolezze che non gli consentono di affrontare le difficoltà di tutti i malati calabresi. Il giudizio sul commissariamento non può che essere negativo. I commissariamenti, specialmente in un settore delicato come quello sanitario, hanno un senso solo se sono provvisori e preordinati a processi di riforma e sviluppo e invece, nel corso degli anni, non si è assistito a niente di tutto ciò. I vari commissari sono stati espressione di lottizzazioni partitiche, orientate non dal manuale Cencelli, che pure aveva una logica, ma da logiche di potere per il potere, alimentate da partitini e partitoni che fanno dell'incoerenza la loro cifra naturale. *(Applausi)*. Il risultato di tutto ciò è sotto gli occhi di tutti: commissari con scarsa, se non nulla, conoscenza del proprio ruolo, che hanno involontariamente tentato di trasformare la tragedia in corso in commedia all'italiana. Ci sono i morti, quelli del Covid e quelli di un sistema sanitario e ospedaliero ormai in ginocchio, a ricordarci che purtroppo non si tratta di una commedia, ma assolutamente di una tragedia. Eppure il Governo, a distanza di un anno dal precedente decreto Calabria, ha deciso di insistere e di rinnovare per altri due anni uno strumento che ha già dimostrato di essere fallimentare. Siamo di fronte a un clamoroso paradosso: è come se si decidesse di curare una persona che ha ingerito del veleno con altro veleno. È questo che sta succedendo adesso in Calabria e adesso la responsabilità è tutta vostra. Non vi è bastato lo squallido teatrino dei tanti commissari da voi nominati, che hanno rappresentato la sanità in Calabria; al Governo non è bastata la manifesta inconsistenza e/o incapacità del generale Cotticelli, da voi nominato, che non sapeva di dover presentare il piano Covid; non gli è bastato il negazionista Zuccatelli, anche lui da voi nominato, che minimizzava circa l'uso della mascherina. Non gli è bastata nemmeno la ridicola giostra di nomi da voi messa in scena, che si è susseguita per circa un mese, con i cittadini calabresi sbigottiti, come se non bastassero la paura e i timori legati all'emergenza da Covid e non solo. Finalmente il Governo, litigioso anche quando c'è da parlare della salute pubblica, ha trovato un compromesso sul nome dell'attuale commissario Longo.

che ha dato lustro alle nostre istituzioni. Si prosegue però, purtroppo, sulla strada erroneamente intrapresa anni e anni fa: Longo non ha le competenze necessarie per amministrare un settore delicato come quello della sanità. *(Applausi)*. La sanità è troppo complicata per essere affidata a gente che di sanità non conosce nulla. Purtroppo la nomina di Longo è frutto dell'ormai storico pregiudizio nei confronti della Calabria, quello stesso pregiudizio per il quale la Calabria non è una questione sociale, politica ed economica, ma resta soltanto una questione criminale le questioni criminali devono essere risolte obbligatoriamente con l'ausilio delle forze dell'ordine. In effetti, ormai, negli ultimi anni in Calabria non si contano più le nomine di ex generali dei Carabinieri o della Guardia di finanza ai vertici delle istituzioni regionali. Ora abbiamo un ex poliziotto alla sanità, come se non fosse bastato l'ex generale Cotticelli. Eppure, quanto è avvenuto negli ultimi mesi in Calabria ha dimostrato che il disastro della sanità e la responsabilità dello sfacelo della sanità non è dei calabresi, né della classe politica calabrese, ma dei commissari nominati da dieci anni a questa parte dal Governo nazionale un Governo che, come ho detto prima, ha rinnovato una formula amministrativa inventata dall'ex ministro Grillo, quando ha presentato il famigerato primo decreto Calabria. Noi di Forza Italia siamo quindi assolutamente contrari a questo decreto-legge. Così come aveva chiesto Jole Santelli, che saluto e abbraccio in qualsiasi parte sia adesso

l'onestà intellettuale che lo ha contraddistinto. Non avete messo mano alle sperequazioni. La cosa più importante è che la Calabria, anche dal punto di vista economico, dev'essere trattata come tutte le altre Regioni d'Italia invece continuate a non considerare questo aspetto. In Calabria non c'è solo bisogno di legalità; la legalità dev'essere accompagnata dalle competenze in materia, quelle che anche questa volta ci avete negato

in nome di quella sempre tanto invocata - e nella sostanza sempre rifiutata - collaborazione istituzionale tra maggioranza e opposizione per il superamento delle carenze più rilevanti di un provvedimento che, non avendo nulla di ideologico, poteva essere occasione ideale ideale per accogliere il nostro contributo di portata strategica e programmatica per la costruzione della strada maestra idonea a traghettare la sanità della Calabria dall'arretratezza - causata da oltre dieci anni di commissariamenti - al futuro, cambio di paradigma irrealizzabile, se non si investe in formazione specialistica multidisciplinare in grado di frenare la mobilità sanitaria dei cittadini calabresi anche per semplici interventi ordinari verso Regioni di confine e non solo nell'area oncologica e dell'elevata complessità.

senza dotarsi dei necessari supporti tecnologici e formativi - da qui l'esigenza del *second opinion* *supporting* specialistico e della telemedicina e senza superare l'imbuto formativo con i nuovi modelli contrattuali di formazione e di praticantato specialistico, non si otterranno mai i risultati che nelle intenzioni vengono dichiarati. È di tutta evidenza che solo il combinato disposto formativo e assistenziale, con investimenti mirati in adeguamento tecnologico, giovani leve, valorizzazione delle competenze e delle conoscenze in un sistema di *second opinion supporting-teaching hospital* e con una rete formativa aperta anche alle strutture non universitarie, può concretamente e in tempi ragionevoli colmare il divario tra lo stato attuale e quanto necessario per la tutela dei diritti di salute dei cittadini calabresi in Calabria i disagi di trasferte sanitarie che, oltre ad essere costose, sono anche ansiogene. L'emendamento 6.0.1, da noi promosso, avrebbe dato l'avvio a questo processo riformatore che avrebbe previsto l'utilizzo degli ospedali di alta specialità, di ricerca a missione traslazionale nell'ambito della biomedicina, andando a concretizzare quel concetto di sussidiarietà solidale in sanità

scientifico (IRCCS) nella diagnosi di qualità e nella continuità terapeutica ad elevato grado di competenza, secondo il modello del *virtual hospital* per le cure croniche integrato capillarmente, a servizio e supporto di contesti profondamente critici come la Calabria e per il rilancio di tutto il Servizio sanitario nazionale a costi attualizzati, dando di più e spendendo di meno. Vale a dire: investire in formazione, innovazione e tecnologia, a garanzia di sostenibilità in chiave universalistica del nostro sistema sanitario nazionale e non solo assunzioni indifferenziate. Ma l'idea di recepire qualcosa che provenga dalle opposizioni, sia pur condiviso nella sostanza, evidentemente non fa parte del vostro modo di interpretare la missione istituzionale incuranti del fatto che non state facendo uno sgarbo all'opposizione, ma state facendo il male della Calabria e dell'Italia tutta.

È evidente a tutti quanto tortuoso sia stato il percorso che ha portato alla nomina del nuovo commissario alla sanità regionale. Non possiamo nasconderlo, onorevoli colleghi: il rinnovo della gestione commissariale è stata una scelta sofferta e difficile, ma ancora necessaria per affrontare una situazione realmente extra-ordinaria, nel senso pieno del termine. Non si tratta di ordinaria amministrazione; non si tratta di rivedere in qualche modo i registri della contabilità (che peraltro, nella ASP cui appartengo, è stata orale per molti anni); non si tratta di riordinare qualche ufficio; si tratta di affrontare lo scandalo degli ospedali iniziati e mai conclusi, di forniture pagate due o più volte (come svelato da inchieste recenti, giornalistiche e giudiziarie), di reparti chiusi a causa di tagli finanziari che riguardano altri Governi, non certo il nostro, ma di chi ha parlato poco fa ed è oggi fra i banchi dell'opposizione. *(Applausi)*. Quindi non accetto lezioni di politica da costoro. Ed è così che in Calabria il primo commissariamento nacque proprio con il governatore di Forza Italia Scopelliti nel 2010; ed è così che in Calabria adesso, siamo all'undicesimo anno, si è reso necessario prorogare questo commissariamento. In Calabria curarsi rischia di diventare un lusso, se non lo è già per alcuni, o addirittura un lucroso affare per altri. Questo, ancora una volta, rende necessario il commissariamento. Ciò ha contribuito a creare un circolo vizioso, per cui i cittadini calabresi, per necessità o per sfiducia, si rivolgono per le ad altre Regioni che dovranno poi ricevere un cospicuo rimborso dal Servizio sanitario regionale calabrese, già drammaticamente indebitato. Si tratta di oltre 300 milioni di euro l'anno di mobilità passiva di soldi dei calabresi ad altre Regioni, che potrebbero e dovrebbero servire per i calabresi. Perché non utilizzare questi soldi (ecco la sfida) per migliorare le prestazioni e curarsi in Calabria? Non è un'operazione facile, lo so: non sarà un'operazione facile, lo sappiamo tutti. Ma dobbiamo metterci tutto il nostro impegno per portare a termine questo fine; non sarà certamente l'intervento salvifico di un uomo solo al comando, di un commissario straordinario, di un magistrato o di una qualunque figura istituzionale, sia pure alta, a sanare, da solo, la situazione drammaticamente difficile della mia Regione. Per questo motivo è necessario che il commissario, come il decreto-legge Calabria-*bis* prevede, sia messo in condizione di circondarsi di un gruppo di collaboratori e di creare un proprio *staff*. Questo prevede il decreto-legge che ci apprestiamo a votare, perché permette al al commissario di avvalersi del supporto di Agenas (fino a 25 collaboratori), così come della possibilità di servirsi della collaborazione della Guardia di finanza, nonché dell'Agenzia delle entrate. Tutti elementi positivi, per cui mi chiedo come mai qualcuno decida di non votarlo. Sarà un percorso lungo, difficile, forse anche pericoloso per gli interessi che andrà per forza di cose a toccare. Ma è un percorso necessario, cari colleghi, e obbligato, per restituire alla mia terra dignità e diritto costituzionale alla cura.

nonostante tutto e nonostante la politica. Si tratta di lavoratori che, anche fuori da ogni gratificazione amministrativa o di carriera, hanno mantenuto e mantengono tuttora in piedi quello che ancora di buono in piedi quello che ancora di buono offre il servizio sanitario regionale calabrese. Uomini e donne di buona volontà, che fanno il proprio dovere semplicemente perché è giusto farlo. Prima di ogni ulteriore considerazione, cari colleghi, tutti noi però dovremmo innanzitutto ricordarci di quelli che hanno tenuto in piedi, come meglio potevano, questo Sistema sanitario regionale. Sì, perché la politica in passato è stata assente nella garanzia dell'assistenza, ma è stata presente dove non doveva: nell'assegnazione delle nomine. Per questo ogni intervento della politica, quella a cui mi piace appartenere, deve iniziare innanzitutto con una richiesta di scuse: scuse per non esserci stata; scuse per aver permesso che tutto ciò accadesse; scuse per non essere stata efficace. Adesso bisogna invertire la rotta. La nomina del commissario Guido Longo non è certamente la conclusione bensì l'inizio di un percorso nuovo, che dovrà portare alla restaurazione di fatto di un sistema sanitario regionale degno di questo nome. Sarà un percorso lungo, come ho detto, e probabilmente non mancherà chi cercherà di sabotarlo, per mantenere il vantaggio del proprio *status quo*, ma questo percorso deve iniziare ora, subito e, cari colleghi, dovrà proseguire come obiettivo di medio termine, al di là dell'orientamento politico di chi governa o di chi governerà la Regione, come come ho già detto nel mio precedente intervento in quest'Aula, con un supporto costante del Governo, che vada anche oltre la vita di questa legislatura, se necessario. Il Governo non si è tirato indietro, demandando ad un commissario la soluzione, unica e straordinaria, di un'emergenza tanto grave. Infatti, all'articolo 7 è previsto che il commissario invii ogni sei mesi una relazione sullo stato di attuazione delle proprie misure al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Presidente della Regione. Questa sinergia dovrà insegnarci molto e dovrà essere una condizione condivisa da tutti, dai politici di oggi e di domani, perché i cittadini da curare non sono dell'uno o dell'altro schieramento, ma bisognosi di cure e basta. In quanto tali, la politica che li rappresenta deve garantire loro una giusta possibilità di curarsi all'interno della propria Regione. C'è di più, cari colleghi: all'articolo 6 vi è anche il contributo di solidarietà per il Servizio sanitario regionale, per il triennio 2021-2023, condizionato però alla presentazione e all'approvazione del programma operativo di prosecuzione del piano di rientro. Questa è un'altra ottima notizia, ma non è solo una questione di fondi, colleghi, perché bisognerà spendere bene. Non si tratta solamente di destinare maggiore denaro a uno specifico sistema sanitario regionale, ma di ricostruire un intero corpo amministrativo, un sistema che permetta innanzitutto una rendicontazione efficace e veritiera dei fondi spesi e dei rimborsi ai servizi. Il tempo della contabilità orale è finito: lo dico in quest'Aula, affinché tutti ascoltino bene, anche dalle mie parti. Onorevoli colleghi, nel pieno della pandemia non è poi ammissibile né accettabile che ci siano interi presidi ospedalieri incompleti o vuoti, perché mai collaudati, mentre c'è chi pensa di costruirne altri.

Eppure, i cittadini calabresi non possono più aspettare: hanno già aspettato tanto, troppo, e chi non ha potuto farlo è andato via. Per questo motivo, interveniamo da subito, con il decreto-legge in esame, con le assunzioni in deroga del personale medico, sanitario e socio-sanitario. L'emergenza amministrativa non può e non deve far passare in secondo piano quella sanitaria. Così, mentre da un lato si mette mano alla gestione finanziaria, dall'altro non aspettiamo oltre e da subito mettiamo in campo forze ed energie nuove, che possano sostenere la popolazione in questo momento difficile e che dovranno essere il personale sul quale ricostruire la nuova assistenza sanitaria regionale.

La gente comune in corsia non incontrerà il commissario regionale, ma dovrà trovare un infermiere nuovo, dovrà vedere un cardiologo in più o un consultorio che aggiunge un giorno di ricevimento, perché è stato aggiunto un nuovo assistente sanitario. Questo dovrà vedere la gente e questo è il nuovo che dovranno riscontrare i cittadini rispetto alle gestioni passate. Questo, solo questo, darà alle persone la percezione di una vera inversione di rotta: non i nostri *slogan*, non le nostre promesse, non le nostre dichiarazioni, ma i fatti. Per questi fatti saremo giudicati e non per quello che avremo detto.

quella che invoco in quest'Aula, come rappresentante dei cittadini di questa terra, è una semplice e rivoluzionaria normalità; la Calabria ha bisogno di quotidiana normalità. Mi avvio a concludere e ringrazio il signor Presidente per avermi concesso un minuto di tempo in più. Per raggiungere questo obiettivo, non potranno esserci mezze misure o compromessi, non più: per questo, con l'articolo 4 abbiamo anche concesso il potere di scioglimento dei singoli enti, in caso di manifesta incapacità gestionale, ma continuando a erogare

dal senso stesso della presenza dello Stato. Sono in gioco, nella mia terra e non solo, giustizia ed equità, perché nel disordine e nel disservizio la malavita e il malaffare prosperano, barattando il diritto con il favore, l'amicizia con il sostegno e la fedeltà con l'ingiustizia. Dunque, insieme alla democrazia è necessario creare una solida

sul contenuto del disegno di legge di bilancio». Ai sensi della predetta disposizione, sul testo approvato dalla Camera dei deputati si procede unicamente ad accertare, sentito il parere della 5a Commissione permanente e del Governo, se il disegno di legge di bilancio rechi disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente. Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente. «La 5ª Commissione permanente, programmazione economica, bilancio, esaminato, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 e sentito il rappresentante del Governo; premesso che il disegno di legge di bilancio, sulla base di quanto previsto dall'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, non soggiace a una regola di copertura, ma a una regola di equilibrio, per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impegnare da esso risultante deve essere coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica; rilevato che, per quanto concerne i profili finanziari, la relazione tecnica aggiornata reca elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare risultante dal disegno di legge di bilancio con gli obiettivi programmatici, attraverso una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare e programmatico e il conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni programmatico, dalla tavola di raccordo emerge che, in corrispondenza di un saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato pari a circa 194 miliardi nel 2021, circa 155 miliardi nel 2022 e 136 miliardi nel 2023, l'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni si attesta a circa 124 miliardi nel 2021, 87 miliardi nel 2022 e 58 miliardi nel 2023. Tali valori del saldo netto appaiono coerenti sia con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge di bilancio, sia con l'indebitamento netto programmatico risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020, come modificate alla luce degli effetti complessivi della manovra; esprime parere favorevole ritenendo che i valori del saldo netto da finanziare risultanti dal disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 siano coerenti con l'indebitamento netto programmatico risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2020, come modificate alla luce degli effetti complessivi della manovra». apre una nuova finestra"). Alla luce del predetto parere, il disegno di legge n. 2054 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023)

la dottoressa Serafin e il dottor Marini, che, a causa della pandemia, si sta prodigando per aiutare tutti noi. Lo faccio adesso e auguro a tutti loro buon anno!

e provoca una progressiva atrofia della muscolatura striata, fino ad arrivare alla fine alla paralisi dei muscoli respiratori, con conseguente morte dei piccoli pazienti entro i primi anni di vita. Oggi, finalmente, esiste una terapia innovativa in grado di correggere il problema genetico e il cui utilizzo è stato da poco autorizzato anche in Italia. Una terapia molto costosa, ma capace, se iniziata precocemente, di determinare il blocco del processo di atrofia, impedendo, di fatto, l'evoluzione progressiva della malattia, riuscendo a sostituire il gene mancante. Il primo trattamento nel nostro Paese è stato effettuato all'ospedale Santobono su una lattante di sei mesi. Un risultato ottenuto prima di tutto dagli scienziati, dai ricercatori e dai genetisti che, dopo anni di studi e ricerche, sono riusciti a ottenere questo brillante traguardo. La ricerca non conosce confini e deve essere incentivata in ogni Paese, e ovviamente anche nel nostro, promossa e facilitata con provvedimenti adeguati. Essa rappresenta nella realtà il futuro del mondo. Un ringraziamento a tutto il personale sanitario, parasanitario e tecnico dell'azienda ospedaliera Santobono, per il loro impegno costante e la loro alta professionalità. Un grazie anche alla direzione tecnica dell'ospedale, che, con lungimiranza, ha permesso di raggiungere questo importante e innovativo risultato. Così come occorre rimarcare le gravi carenze strutturali e di programmazione nella mia Regione, non si può non sottolineare, con soddisfazione e orgoglio, quanto accaduto perché dimostra il grande lavoro svolto dalle eccellenze professionali e dalle competenze che in essa operano. L'eccezionale lavoro di squadra ha pagato e ha reso possibile un traguardo che, fino a poco tempo fa, sembrava impossibile, coinvolgendo strutture, servizi e personale dell'ospedale pediatrico napoletano. Concludo facendo due considerazioni: da un lato, l'importanza degli *screening* neonatali per una diagnosi precoce, condizione fondamentale, come in questo caso, per un trattamento il più possibile iniziato prima che gli effetti della malattia siano irrecuperabili; dall'altro, in un mondo in cui le politiche sanitarie sono spesso dettate da parametri di *budget* prefissati e da scarsa disponibilità, poter salvare una vita umana non deve essere assolutamente legato a un costo economico, pur altissimo che sia, come nel caso della piccola paziente. Speriamo che per le tante altre malattie genetiche, purtroppo ancora senza terapia risolutiva, la ricerca possa riuscire, come per la SMA, a far intravedere la luce tanto attesa alla fine del *tunnel*.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, a settantacinque anni dalla nascita dello Statuto speciale siciliano e a venti dalla cosiddetta riforma federalista, la Regione Sicilia attende ancora i propri decreti attuativi. Questi, in verità, ad oggi ci sono, ma in genere non sono in armonia con i dettami statutari; e quando non lo sono, sono violati persino da legge ordinaria. Quanto accaduto con l'ultima legge di bilancio dello Stato, che ha assorbito incostituzionalmente in Agenzia delle entrate la società Riscossione Sicilia, mentre lo Statuto e i decreti attuativi dispongono diversamente, rappresenta un'ennesima illiceità ai danni dei siciliani. A dispetto di una vulgata sparsa ad arte, la realtà è che oggi la Regione e i Comuni che da questa dipendono hanno già la totale autonomia solo dal lato delle spese, poiché assolvono a quasi tutte le funzioni, mentre le entrate sono saldamente nelle mani dello Stato. Tranne che per polizia, carceri e insegnanti, i siciliani pagano già tutto da sé, mentre solo una frazione non proporzionale di tributi è loro attribuita. Dopo decenni di abusi già denunciati nella scorsa legislatura regionale siciliana durante il governo Crocetta, questi, anziché porvi rimedio, ha firmato accordi capestro in cui le illegalità venivano sanate rendendo legale ciò che era e rimane illegale, incostituzionale e insostenibile. In queste condizioni e con la catastrofe pandemica, i bilanci non si possono più chiudere, e - si badi - non per eccesso di spese, ma perché le entrate naturali della Regione sono dirottate altrove.

Si parla di insularità anche nell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che significa anche fiscalità di vantaggio secondo la tendenza delle Azzorre. Altra violazione riguarda la mancata esitazione di una legge regionale siciliana votata all'unanimità dalla deputazione tutta, relativa all'istituzione delle zone franche montane. Sono 132 i Sono 132 i Comuni coinvolti e da diciotto giorni dei loro rappresentanti manifestano in contrada Irosa, lungo la Palermo-Catania, per chiedere il completamento dell'*iter* legislativo. Il Senato sta contravvenendo agli articoli 73 e 74 del Regolamento. Chiedo pertanto che, entro le prossime due settimane, si concluda l'*iter* qui in Senato per dare ristoro alle famiglie e alle piccole e medie imprese del territorio colpite dal Covid, e non solo. Diversamente, avremo un motivo in più per ricorrere alla Corte di giustizia europea. **Atti